Grazie, Presidente. in relazione al quesito sollevato in tema di tetto reddituale in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta quanto segue. Va intanto ribadito quanto già indicato in data 22 marzo 2023 alla Camera dei deputati, in sede di risposta all'interrogazione 5-00556. Pertanto, si rammenta che il decreto interdirigenziale in questione, sottoscritto dalla preposta articolazione ministeriale e dal Ragioniere generale dello Stato, del 3 febbraio 2023, segue il precedente emanato in data 23 luglio 2020, con il quale si era tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018, ragion per cui, in una logica di continuità temporale con il precedente, è riferito al periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020. Il Ministero, inoltre, alla luce della significativa variazione in aumento dell'indice dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il biennio 1° luglio 2020 - 30 giugno 2022, pari al 9,4 in base ai dati acquisiti dall'Istituto nazionale di statistica, ha immediatamente avviato le opportune interlocuzioni per l'emanazione di un nuovo decreto che tenesse conto degli effetti sopra descritti. Conseguentemente, con recentissimo decreto

12.838,01. Il provvedimento è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 giugno del 2023. Quanto sopra evidenzia la doverosa attenzione che il Ministero assegna alla tematica, certamente assai delicata poiché inerente all'effettività del diritto di difesa dei non abbienti, categoria vulnerabile e quindi vieppiù meritevole di tutela. È doveroso, infine, riferire che il tempestivo intervento ministeriale ha ricevuto il gradito plauso del Consiglio nazionale forense, ente esponenziale

dovendo intervenire, come disposto per legge, all'adeguamento con riferimento al biennio precedente, si è invece fatto riferimento al biennio ancora precedente, quindi c'è stato un clamoroso errore di disattenzione, ancora più clamoroso perché riguarda l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, perché il gratuito portoncino riguarda la difesa dei non abbienti e quindi una fascia di popolazione piuttosto ampia che si trovava comunque ancora impossibilitata ad accedere alla garanzia del diritto di difesa. Avevo presentato un'interrogazione successivamente a febbraio e dopo la mia interrogazione, che ovviamente raccoglieva l'inquietudine di tutta l'avvocatura associata e non solo, a maggio il Governo è stato costretto a intervenire su se stesso. lieta che sia stato corretto l'errore, ma non possiamo che sottolineare una disattenzione, ancora una volta, verso i meno abbienti e verso l'effettività dell'esercizio

di chi in questo momento si trova in condizioni reddituali particolarmente basse, come vediamo, coinvolgono tantissimi diritti primari, perché prima c'è il diritto

risultano aver avuto una recente evoluzione positiva. Secondo quanto emerso in esito al confronto di fine settembre tra le rappresentanze sindacali e i vertici aziendali, infatti, l'azienda ha dato rassicurazioni sulla situazione produttiva dello stabilimento per il quale si prospetta un incremento

Di conseguenza, i vertici aziendali hanno stabilito di sospendere i contratti di solidarietà del personale da tempo in essere. Ciò premesso, resta alta l'attenzione del Governo verso l'importante e storico gruppo Marelli. Anche in questa occasione tengo a ricordare come, all'emergere per esempio di criticità presso lo stabilimento Marelli Europe di Crevalcore (Bologna), è stato tempestivamente chiamato presso il MIMIT un tavolo di crisi volto ad affrontare le problematiche dell'azienda, con i possibili risvolti occupazionali. Il primo incontro del citato tavolo si è tenuto il 3 ottobre scorso e un nuovo incontro è già programmato per il prossimo 8 novembre. Sebbene l'incontro del 3 ottobre fosse dedicato prevalentemente alle sorti del citato stabilimento di Crevalcore, in quell'occasione il ministro Urso ha chiesto al gruppo di presentare un piano industriale con le previsioni produttive ed occupazionali di lungo periodo di tutte le sedi del gruppo Marelli in Italia. Infatti, tra le priorità di questo Governo vi è quella di accompagnare il complessivo rilancio della produzione dell'intero settore *automotive*,ivi compresi gli importanti stabilimenti del gruppo Marelli, che in Abruzzo, come del resto per l'intero Paese, rappresentano una rilevante risorsa economica e occupazionale. Senza dubbio - come ricordato in una delle interrogazioni in parola - su tale settore ha influito la nascita del gruppo Stellantis, avvenuta nel gennaio 2021 con la fusione dei gruppi Fiat Chrysler (FCA) e PSA. Sulla vicenda Stellantis, tuttavia, voglio ricordare l'impegno profuso dal Governo, che ha inteso recuperare un dialogo, completamente mancato nel passato, con il medesimo gruppo e con tutti gli *stakeholder* del settore. Il Governo si muove quindi con una visione e una strategia di sistema, ma al contempo non intende lasciare irrisolte le problematiche specifiche sotto il profilo produttivo e occupazionale degli attori coinvolti nella filiera, come dimostra la pronta convocazione del tavolo innanzi richiamato. Quest'ultimo potrà quindi costituire una sede di confronto rispetto ai diversi siti produttivi del gruppo Marelli, qualora se ne ravvisasse la necessità, fermo restando che ad oggi la situazione dello stabilimento di Sulmona appare rassicurata e presidiata dal confronto tra le parti tenuto a livello aziendale.

per l'economia abruzzese, il gruppo Marelli rappresenta - come ha detto - una realtà aziendale di assoluta importanza. Le difficoltà del comparto tuttavia ricadono anche sulla realtà industriale della Marelli, generando pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali. Come già detto, l'azienda ha comunicato l'intenzione di considerare, per lo stabilimento di Sulmona, 100 esuberi nel 2024, dopo averne dichiarati precedentemente 135; un sensibile contenimento il cui ottimismo traspare anche dalle sue parole - che fa il paio con la chiusura del contratto di solidarietà, ma che ovviamente non può e non deve lasciare tranquilli. Né possono ritenersi rassicuranti le notizie di stampa, che proprio in questi giorni rilevano l'assunzione di personale interinale ad integrazione dei lavoratori in forze nello stabilimento sulmonese. Questi dati apparentemente positivi sono determinati in realtà da periodi di recupero che - come ha detto - il gruppo Stellantis ha attivato nei mesi alle nostre spalle e che hanno dunque determinato risparmi e contenimento delle risorse. Né può rassicurare, in tutta onestà, Sottosegretaria, la notizia di presunte nuove produzioni in cui dovrebbe essere impegnato lo stabilimento di Sulmona, in merito alle quali non vi è ancora chiarezza e soprattutto non vi sono indicazioni di dettaglio sulle risorse di personale da dedicarvi. peraltro sconterebbero la grave carenza di manutenzione dello stabilimento peligno, senza un efficace programma di investimenti straordinari, dei quali non si ha alcuna notizia. Una situazione, dunque, che resta nel suo complesso preoccupante e che esige da tempo un intervento più deciso del Governo. Di fronte a questa urgenza,

alla crisi del gruppo industriale, come appena descritta, per la quale l'azienda ha dichiarato di voler confermare, anche per il 2024, l'istituto del contratto di solidarietà. Nel sito industriale di Sulmona lavorano 490 persone: professionalità e famiglie che non vedono di fronte una prospettiva chiara. La produzione di forniture per lo stabilimento Stellantis di Atessa ha subìto pesanti contrazioni, dettate da una revisione delle strategie aziendali di questo importante gruppo. A questo si aggiunga che la fornitura di semiconduttori ha subìto un sensibile rallentamento durante il periodo della pandemia; ciò non ha consentito una produzione completa e ha contribuito a una condizione di generale incertezza del settore *automotive*. Di fronte a tutto ciò, le forze sociali e sindacali hanno tenuto alta l'attenzione e alimentato un ampio livello di mobilitazione. Le voglio ricordare che, nel corso dello sciopero dello scorso 10 luglio, ho avuto modo di ascoltare personalmente le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori; ero ai cancelli della fabbrica a Sulmona non c'erano parlamentari di maggioranza né c'era il Governo. Quindi do un sommesso consiglio: stare ai cancelli con lavoratrici e lavoratori quando ci sono scioperi e provare a interloquire di fronte alle preoccupazioni aiuta anche a governare e a legiferare meglio. Abbiamo il dovere di seguire questa vertenza con il massimo impegno e pretendiamo dal Governo un'attenzione concreta, capace di tutelare i posti di lavoro e la produttività di un settore fondamentale per il Paese e per il territorio. Insoddisfatti di come oggi in quest'Aula sia stato affrontato il tema, assicuriamo a tutti i portatori di interessi che continueremo a tenere alta l'attenzione, convinti che siamo nell'ambito della transizione ecologica. Le istituzioni hanno il dovere di accompagnare ognuno e non lasciare nessuno indietro: queste sono parole che ho sentito anche dalla presidente Meloni, ma di fronte a queste c'è bisogno davvero di una strategia più complessiva, di una politica industriale della quale discutere anche in Parlamento. Occorrono pertanto non solo tavoli di crisi, che pure sono necessari, ma anche capire esattamente come noi non lasciamo nessuno indietro, accompagniamo la transizione digitale ed ecologica e facciamo sì che ogni lavoratrice e ogni lavoratore - in carne ed ossa, non ridotti a numeri - possano passare da una all'altra condizione, da un modello di sviluppo all'altro. Questo è davvero il tempo per affrontare una discussione del genere, perché abbiamo bisogno di una politica economica che affronti questo tempo e non di rinvii o denunce di complotti. Abbiamo bisogno di capire esattamente come cambiamo la produzione e come facciamo sì che questo non significhi perdita di posti di lavoro, ma se mai miglioramento di posti di lavoro, accompagnamento, ammortizzatori, nuove strategie. Ecco, su questo abbiamo bisogno di fare una discussione più profonda che poi si cali anche in territori come quelli che riguardano l'interrogazione odierna: Sulmona, l'Abruzzo, la Magneti Marelli, l'*automotive*.

e poco ci dice su quelle che saranno le prospettive future dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. Prima che in quest'Aula, infatti, la risposta l'abbiamo letta sui giornali: abbiamo letto che l'azienda è tornata indietro su alcune decisioni che aveva preso poc'anzi e di questo ne siamo felici. Non è chiaro quale sia stato il contributo del Governo per la risoluzione di tali questioni. Di certo, la mobilitazione degli operai e delle sigle sindacali ha portato i propri frutti. in Abruzzo dà lavoro a 25.000 persone; in particolare, i dipendenti della Marelli sono 550, più tutto l'indotto che le viene creato intorno. La domanda è sul futuro

Sull'operato della Regione Abruzzo stendo un velo pietoso: non si è vista la presenza di un ente regionale che avrebbe dovuto esercitare la sua tutela o comunque interessarsi alle questioni che spesso sono state sollevate e per le quali è stata richiesta l'attenzione dello stesso Presidente della Regione. Parliamoci chiaramente: quello che quello che vogliamo scongiurare è una situazione simile a quella di Crevalcore, che aveva delle commesse contrattualizzate fino al 2028; un'azienda che è stata chiusa improvvisamente per le scelte dei vertici di Stellantis. Anzi, vorrei vorrei esprimere tutta la vicinanza mia e del MoVimento 5 stelle a questi lavoratori e a tutti coloro che lottano per il diritto al proprio lavoro. Per Sulmona ci aspettiamo delle risposte e dei fatti concreti. Un Paese civile, signora Sottosegretaria, non può dire loro: state tranquilli fino a dicembre e poi si vedrà. Chiedo a lei e al Governo di monitorare con maggiore attenzione tutte le situazioni che si rifanno al sito Magneti Marelli di Sulmona e di pianificare, per quanto sia possibile, delle strategie future che tengano conto di tutte le variabili che sono in campo. Questo lo dobbiamo e lo dovete agli operai e a tutte le loro famiglie.

Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti per il quesito. La rilevanza tecnologica della società Comau e il ruolo di primo piano che essa svolge nel mercato dell'automazione industriale sono ben conosciuti al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Proprio per tali sue specifiche caratteristiche, la società è anche coinvolta in importanti iniziative sostenute dal Ministero. Comau, infatti, è *partner* e socio fondatore del MADE - Competence Center*,* creato con il sostegno e su iniziativa del MIMIT per avvicinare le imprese italiane all'Industria 4.0, realizzando, a tal fine, attività di orientamento, formazione e supporto per la realizzazione di progetti di innovazione. Nel recente passato, con il Governo Draghi e il ministro Giorgetti, il MIMIT ha inoltre autorizzato la stipula di un accordo per l'innovazione, relativo ad un investimento complessivo di diciotto milioni di euro, con le Regioni Lombardia e Sicilia, le aziende ST Microelectronics e FCA Italy*,* oltre che con Comau, naturalmente, per la realizzazione di un progetto innovativo nel settore delle produzioni microelettroniche. D'altra parte, però, Comau è una società del gruppo Stellantis e, come tale, le vicende che la riguardano esigono di essere considerate nell'ambito più ampio, che vede tuttavia il Governo fortemente impegnato fin dal primo giorno. È noto, infatti, che nell'assenza, purtroppo, di iniziative poste essere negli anni passati, il Governo ha dovuto recuperare un dialogo con il gruppo Stellantis, che è tuttora costante, costruttivo e attento alle dinamiche dell'intera filiera e che intende giungere ad un piano di lavoro condiviso, per il miglioramento della competitività e della produttività dell'industria *automotive* nazionale. Vi è, pertanto, piena considerazione, in questo contesto di raffronto e di condivisione, per tutti gli attori del settore e ciò a prescindere anche dalle possibilità offerte dall'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, che richiedono precisi presupposti, ma che al momento non risultano concretizzati. Per quanto riguarda la preoccupazione che la costituzione di un eventuale *spin off* possa indebolire Comau, con conseguenti impatti negativi sull'occupazione,

Noi parliamo di un'azienda sana, con 700 dipendenti, con una crescita degli ordini, anche soltanto in questo ultimo anno, di oltre il Un'azienda assolutamente rinomata, importante sui mercati internazionali, ma che non solo non ha aumentato il numero dei dipendenti, ma lo ha quasi dimezzato; con tre anni di ritardo nella presentazione di un piano industriale, più volte chiesto, più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali, in rappresentanza ovviamente dei

Si paventa continuamente questa volontà di FCA, oggi Stellantis, di attuare un'ulteriore *spin-off*, come ha fatto anche, per la verità, in altre situazioni. Penso ad esempio alla scelta su Iveco, che comunque ha avuto risultati positivi,

non giustifica assolutamente la mancanza totale di assunzioni, anzi quasi un dimezzamento del personale. Questi articoli continui sui giornali, con posizioni sempre più ambigue da parte della proprietà sullo *spin-off*, creano condizioni di grande grande allarme e preoccupazione tra i lavoratori e non solo.

Perché questo è un messaggio che è trapelato anche in alcune parole del Ministro, ma che rimangono sempre notizie non definite. ringrazio per la risposta, ma sarà comunque necessaria da subito una convocazione al Ministero tra le parti sociali e l'azienda, perché si faccia finalmente chiarezza e si capisca quali sono le prospettive di un'azienda che sta crescendo. Non parliamo di un'azienda in crisi, ma di un'azienda che sta crescendo, ma che contemporaneamente dimezza il personale, non presenta piani industriali e continua ad aleggiare l'ipotesi di uno *spin-off* di cui non si sa altro.

Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti dato che il tema è oggettivamente delicato. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere evidenziato che, sulla scorta del contenuto della nota estesa dalla presidenza della Corte di appello di Roma, la vicenda in esame può essere così ricostruita nei suoi punti focali. L'avvocato in questione, nel corso di un processo celebrato innanzi alla seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale, chiedeva il rinvio per legittimo impedimento dell'udienza, fissata per il 14 aprile 2023, a causa dell'esposta necessità di accompagnare il figlio di due anni ad effettuare un esame diagnostico all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma in regime di *day hospital*. L'avvocato in questione, con riferimento all'udienza fissata per il 14 aprile 2023, nominava una sua collega quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 102 del codice di rito penale. La seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale rigettava l'istanza di rinvio presentata dall'avvocato, con riferimento all'udienza fissata per il 14 aprile, perché non tempestiva e non adeguatamente motivata in relazione al carattere assoluto dell'impedimento dedotto. La decisione adottata dalla II sezione penale del tribunale di Roma, in composizione collegiale, appare conforme alla vigente disposizione normativa di cui all'articolo 420-*ter*, comma 5, del codice di procedura penale e agli insegnamenti in materia della Corte di cassazione, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di differimento, è necessaria non solo la tempestiva prospettazione dell'impedimento, ma anche l'indicazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura penale. L'istanza di rinvio deve essere considerata tempestiva se viene presentata prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza dell'impedimento, elemento questo che va ritenuto insussistente nel caso di specie, posto che la richiesta di rinvio veniva trasmessa dall'avvocato in questione alla cancelleria della II sezione penale del tribunale di Roma solo in data 12 aprile 2023, alle ore 18,48, a fronte di un impedimento determinato da ragioni familiari, conosciuto dal difensore istante sin dal 28 marzo 2023. La richiesta di rinvio avanzata in data 12 aprile 2023 dall'avvocato in questione non può comunque ritenersi adeguatamente motivata in relazione al carattere assoluto dell'impedimento addotto (questo a normativa vigente), visto che, anche in considerazione della parificazione a livello normativo dei diritti e dei doveri di entrambi i genitori nella cura e nell'accudimento dei figli minori, il difensore aveva l'onere di dimostrare l'eventuale impossibilità dell'altro genitore di accudire idoneamente il figlio in occasione del su indicato esame diagnostico. Nell'udienza celebrata il 14 aprile la II sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale, con apprezzabile spirito di collaborazione, prima di adottare il provvedimento formale di rigetto dell'istanza di rinvio, avanzata il 12 aprile dallo stesso avvocato, tentava, senza esito positivo, di fare contattare dal sostituto processuale il difensore istante. Pertanto, in questo contesto e con quegli orientamenti giurisprudenziali, non rilevandosi anomalie processuali dei magistrati del tribunale di Roma che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, deve concludersi nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio di iniziative segnatamente di carattere ispettivo spettanti al Ministero della giustizia. si fa presente che il tema, indubbiamente sensibile, è all'attenzione del Parlamento; sul piano generale il Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2023 ha approvato un disegno di legge, poi trasmesso all'esame del Parlamento il 20 luglio, volto ad ampliare e rafforzare il diritto di difesa degli indagati, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, sin dall'avviso di procedimento penale. Nello specifico si segnala che presso la Commissione giustizia del Senato è incardinato e risultano svolte numerose audizioni, il 729 del 2023 che prevede la modifica dell'articolo 420-*ter,* comma 5, del codice di procedura penale, individuando quale legittimo impedimento del difensore il proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute.

Credo che chiunque di noi, donna e lavoratrice, si sia trovata nella propria esperienza di vita in situazioni in cui ha sentito fino in fondo, sulla propria pelle, se posso usare questa espressione, la lacerazione tra i doveri, la necessità di accudimento dei propri figli, e la necessità di essere presente nel luogo di lavoro. Non è una lacerazione che riguarda solo le nostre vite personali o una questione privata, ma è un'incapacità dell'organizzazione del lavoro e del *welfare* di questo Paese a sostenere davvero le donne che lavorano. Non è un caso che lo stesso presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento abbia detto: «Dignità è non dover essere lavoro e maternità». Siamo tutti d'accordo e sosteniamo tutti che in questo Paese c'è un problema di denatalità. L'interrogazione, oltre al caso singolo e quindi alla vicenda dell'avvocata che comunque, vorrei sottolineare, ha ricevuto la solidarietà del Consiglio nazionale forense e dello stesso Comune di Roma che ha chiesto un osservatorio sulla questione, apre una discussione più generale su come vogliamo

che poteva esserci in quel caso l'altro genitore, come è stato detto. Nel caso specifico vorrei sottolineare come sia prassi ormai consolidata decidere al momento della celebrazione dell'udienza, prescindendo dal momento in cui è stata depositata l'istanza, se la stessa venga rimandata per rimandata per legittimo impedimento. L'altra avvocata era stata indicata proprio per poter capire se l'udienza veniva rimandata. In ogni caso,

Signor Presidente, si tratta di una risposta che contiene un certo numero di dati, che ovviamente poi saranno a disposizione dell'interrogante, affinché ne abbia diretta contezza, al di là del mio *speech*. Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante, riportata la notizia di una rissa verificatasi il 30 giugno 2023 nel carcere Regina Coeli di Roma, e riferite le criticità, in particolare di organico, rilevabili in detto carcere, avanza quesiti sulle iniziative che si intendano perciò assumere. Orbene, come ribadito in occasione di risposte a interrogazioni di analogo tenore, in tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), pone forte attenzione all'esigenza di garantire un efficace *turnover* del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati. riduzione - com'è noto - è stata operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi, che hanno rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del Corpo della polizia penitenziaria, su cui andrà evidentemente reimpostata una politica di forte implementazione. Sul punto, giova evidenziare la ferma volontà di inversione del *trend*, posto che attualmente l'organico totale (42.865 unità) è tale grazie all'incremento di 1.000 unità del ruolo agenti-assistenti disposto con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. ln concreto, tuttavia, il personale del Corpo di polizia penitenziaria amministrato ammonta a 35.960 unità. Va poi rammentato che nell'arco del quinquennio 2021-2025 è autorizzata, oltre al *turnover*, l'assunzione straordinaria di complessive ulteriori 2.804 unità. Quanto alla precipua situazione del carcere di Regina Coeli, si evidenzia che, a fronte di un organico previsto pari a 516 unità, ne risultano presenti 321, comprese 135 distaccate in uscita e 50 in entrata, inferiori dunque di 195 unità rispetto a quelle previste. si rilevano nel ruolo dei funzionari (-1), degli ispettori (-7), dei sovrintendenti (-32) e degli agenti-assistenti (-28). Con riferimento alla carenza del ruolo dei funzionari, si rappresenta che è stato conferito l'incarico di comandante di reparto a un primo dirigente di Polizia penitenziaria dall'11 settembre 2023. Circa il ruolo degli ispettori, si evidenzia che, all'esito di procedura concorsuale per complessivi 691 posti, l'organico della casa circondariale di Roma Regina Coeli è stato incremento di dieci unità maschili e che inoltre, all'esito di ulteriore concorso per 411 posti, l'amministrazione terrà nella massima considerazione la situazione del carcere romano, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità per quel Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si evidenzia che, in seguito a concorso interno per complessivi 583 posti, il DAP ha già disposto di assegnare al carcere romano 21 unità maschili e quattro femminili, il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione. Quanto al ruolo di agenti-assistenti, si rappresenta che l'organico è stato incrementato, nell'anno 2022, di 29 unità maschili e due femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso. Ciò riferito, va precisato che le lesioni (frattura della mandibola) occorse all'operatore di polizia non sono collegate ad alcuna rissa tra detenuti, bensì ad altro episodio, verificatosi sempre il 30 giugno 2023, allorquando il detenuto H.F., al termine del colloquio con la propria convivente, senza alcuna ragione apparente, sferrava un pugno all'assistente di Polizia penitenziaria, colpendolo al volto. Per tale fatto il ristretto veniva dapprima sanzionato con quindici giorni di esclusione dalle attività in comune, spostato di sezione, per poi essere trasferito, il 15 luglio 2023, per ragioni di ordine e sicurezza, presso la casa circondariale di Viterbo, nuovo complesso. Gli episodi di violenza tra detenuti menzionati sono invece riconducibili alla mattinata del 25 giugno 2023, allorquando, poco prima dell'inizio delle celebrazioni della santa messa, il detenuto C.G., alla vista di altro detenuto, iniziava a ingiuriarlo con espressioni volgari, provando a colpirlo, altresì, con una delle sedie predisposte per la celebrazione della messa. Ne scaturiva una rissa poiché intervenivano altri detenuti. Il personale riusciva poi a sedare la colluttazione e nei confronti dei detenuti coinvolti veniva disposto il divieto d'incontro. Un'unità di personale intervenuta riportava due giorni di prognosi, a seguito di sospetto strappo muscolare al ginocchio sinistro, mentre un detenuto coinvolto negli scontri veniva inviato in ospedale per frattura di un dito. Per tali disordini, la direzione avviava il procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti individuati quali responsabili degli stessi e li sanzionava con quindici giorni di esclusione dalle attività in comune; provvedeva, poi, a informare l'autorità giudiziaria per gli aspetti penalmente rilevanti della vicenda. Il 26 giugno 2023 quattro dei cinque detenuti suddetti venivano trasferiti, per motivi di ordine e sicurezza, presso altre sedi del distretto. Quanto alle presenze detentive, al 25 luglio 2023, presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli risultavano presenti un totale di 998 detenuti, a fronte di una capienza pari a complessivi 607 posti disponibili, rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari al 164,42 per cento. Relativamente al problema del sovraffollamento, il DAP, oltre a continuare l'attività di riqualificazione del patrimonio edilizio concesso in uso governativo, è da anni impegnato in un programma finalizzato all'aumento del numero dei posti regolamentari mediante il recupero di quanto già disponibile e l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica in complessi esistenti, ovvero realizzando nuovi padiglioni detentivi in comprensori già sedi penitenziarie. La realizzazione di 8 padiglioni dovrà essere necessariamente ultimata entro l'anno 2026 e produrrà, complessivamente, ulteriori 640 posti detentivi. Entro il 2024 dovrebbe essere ultimato, peraltro, il nuovo padiglione da 400 posti in costruzione presso la casa circondariale, nuovo complesso, di Roma Rebibbia. Il completamento dell'anzidetto piano di interventi potrà consentire di contrastare con maggiore adeguatezza ed efficacia la problematica relativa alla condizione di sovraffollamento che affligge il sistema penitenziario, nonché assicurare una maggiore disponibilità di spazi utili il superamento dell'ulteriore criticità legata alla carenza di superfici e ambienti utili per le attività trattamentali. In relazione agli investimenti volti al miglioramento delle condizioni detentive, il preposto DAP sta procedendo all'attuazione di quanto programmato per realizzare un modello di esecuzione penale fondato sull'ampliamento delle opportunità di lavoro professionalizzanti, al fine di migliorare la qualità degli interventi diretti all'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale. In particolare, si segnala che, con la legge di bilancio 2023, sono stati incrementati di due milioni di euro i fondi relativi alla retribuzione del lavoro dei detenuti, passando da euro 121.016.095 nel 2022 euro 123.016.095 nel 2023. La Cassa delle ammende, inoltre, ha finanziato un programma nazionale per l'incremento delle opportunità di lavoro professionalizzanti, per un importo complessivo di 8 milioni di euro, rivolto a 1.500 detenuti. Il Ministero sta poi studiando convenzioni private con Il Ministero sta poi studiando convenzioni private con enti che consentano di incrementare le *chance* lavorative all'interno degli istituti di pena. Continua poi la collaborazione con le Regioni per rafforzare la coesione e la sicurezza sociale. Sono stati approvati dalla cassa delle ammende i programmi per l'inclusione sociale dei detenuti e delle persone sottoposte a misure di comunità, nonché inerenti al sostegno dei rapporti familiari e con i figli minori. Dalla realizzazione dei suddetti programmi la cassa delle ammende prevede il coinvolgimento di 7.638 destinatari, per un investimento complessivo - per il triennio 2023-2025 - di euro 20.662.100, di cui 14 milioni di euro a carico della cassa delle ammende e 6.662.100 e 6.662.100 a carico complessivamente delle Regioni interessate ed in attuazione di quanto previsto nell'atto di indirizzo del Ministro della giustizia e nell'accordo sancito il 28 aprile 2022, tra Governo, Regioni e autonomie locali, nonché del protocollo attuativo stipulato il 28 giugno 2022 tra Ministero della giustizia, Conferenza delle Regioni e Province autonome e cassa delle ammende. Sono stati previsti, altresì, interventi per la prevenzione del rischio suicidario e del disagio psichico in carcere, nonché per migliorare la qualità degli interventi trattamentali destinati ai detenuti stranieri e a coloro che vengono sottoposti a pene sostitutive della detenzione, in modo da assicurare maggiore controllo durante l'esecuzione penale esterna, per euro 3.293.685. Per completezza, si rappresenta, infine, che è stato emanato il decreto interministeriale di riparto del fondo istituito *ad hoc*, con l'articolo 1, comma 856, della legge di bilancio 2023, con il quale sono stati messi a disposizione dei provveditorati regionali 4 milioni di euro per il corrente esercizio finanziario e 5 milioni di euro a regime, proprio per favorire il reinserimento sociale delle persone detenute e di quelle sottoposte a misure penali di comunità, per l'assistenza e la cura dei tossicodipendenti, per la cura e l'assistenza sanitaria e psichiatrica dei detenuti, in collaborazione con le Regioni.

il grande lavoro svolto dal Governo in questo anno su un tema rispetto al quale ovviamente non potevamo e non possiamo immaginare che in un lasso di tempo

- sia per il reinserimento lavorativo, la rieducazione e tutto quello che è necessario. Pochi mesi fa nel carcere di Rebibbia è stato inaugurato un nuovo spazio

la certezza della pena. Il fatto è che chi ha una pena da scontare deve farlo nei tempi e nei modi dovuti,

Cb, SCN))*. Signor Ministro, negli ultimi anni, l'Alto Adige-Südtirol è diventato teatro di frequenti episodi di violenza, anche da parte di minori. Soprattutto Bolzano e Merano sono nella morsa della piccola criminalità, che purtroppo vede spesso coinvolti migranti, sia senza permesso di soggiorno, sia di seconda generazione. Per discutere di tale problema, lo scorso 5 ottobre si è tenuto un vertice nella sede del commissariato del Governo a Bolzano. Dall'incontro è emersa la necessità di più agenti per le strade e maggiori controlli, specialmente nei luoghi più a rischio e durante le ore notturne. A tal fine, gli organici delle Forze di polizia appaiono non solo sottodimensionati, ma anche mal distribuiti sul territorio provinciale: il commissariato di Merano, Comune di 41.000 abitanti, ha 40 agenti a disposizione, lo stesso numero del commissariato di San Candido, Comune di 3.000 abitanti. Anche le Forze di polizia locale, con un totale di 380 agenti su tutto il territorio provinciale, sono sotto organico: stando alle linee guida del Ministero dell'interno, infatti, dovrebbe esserci un agente ogni 1.000 abitanti. Peraltro, da diversi anni la Polizia locale chiede di essere classificata come Forza di polizia "paritaria", il che richiederebbe una modifica dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, al quale solo i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e il Corpo forestale hanno responsabilità di pubblica sicurezza. Infine, sempre in un'ottica di sicurezza, si ritiene ormai indispensabile la costruzione del nuovo carcere di Bolzano: l'attuale struttura carceraria è inadatta, tanto che non sono mancati detenuti che hanno chiesto allo Stato un risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 35-*ter* della legge penitenziaria, perché non è stato loro garantito lo spazio minimo prescritto. Si chiede pertanto di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire prontamente per risolvere il problema relativo al sottorganico delle unità di Polizia in Alto Adige-Südtirol, anche attraverso una migliore distribuzione sul territorio provinciale; se non intenda intervenire sulla legge succitata per equiparare le Forze di polizia locale alle altre Forze di polizia e se non concordi sulla necessità di costruire il più presto possibile un nuovo carcere a Bolzano che sia idoneo a garantire le prescrizioni della legge penitenziaria.

di personale, l'Arma dei carabinieri con una forza effettiva di 818 unità e la Guardia di finanza con 410 militari. Si tratta di numeri che il Governo ha intenzione di incrementare, proseguendo peraltro le politiche assunzionali già avviate con la legge di bilancio per l'anno in corso e che troveranno ulteriori risorse finanziarie in quella per il prossimo anno. La situazione della Provincia di Bolzano è alla costante attenzione del commissario del Governo, che - come ha ricordato l'onorevole interrogante con riferimento al Comune di Merano - in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 5 ottobre scorso ha deciso di incrementare i servizi di controllo del territorio sia ordinari che straordinari, anche con l'ausilio del personale di rinforzo del reparto prevenzione crimine assegnato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Dall'inizio dell'anno al 10 ottobre scorso l'attività di prevenzione e di controllo del territorio nelle città di Bolzano, Bressanone e Merano si è potuta avvalere di rinforzi assegnati a quel territorio, che hanno consentito di realizzare 102 interventi, con l'impiego di 207 equipaggi e 621 unità di personale. Quanto al tema della valorizzazione delle polizie locali, la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale è da tempo interessata da proposte di riforma, anche in questa legislatura, tese a rivedere in modo organico le competenze, le funzioni, i ruoli e le qualifiche del personale della polizia locale, nonché il trattamento economico e previdenziale e il relativo stato giuridico. Il Ministero dell'interno reputa fondamentale dare risposte concrete alle legittime richieste degli operatori della polizia locale e mettere a sistema le esperienze maturate sui territori, che hanno visto la proficua collaborazione tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli amministratori locali. L'obiettivo è quello di introdurre un quadro ordinamentale coerente con i sempre più pregnanti compiti affidati alle polizie locali nella lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i soggetti coinvolti a vario titolo. In questa direzione ho voluto costituire, in seno al mio Ministero, un gruppo di studio sul tema, i cui lavori auspico possano a breve tradursi in un disegno di legge governativo in materia, da sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri. Quanto al riferimento al nuovo carcere di Bolzano, il Ministero della giustizia mi ha comunicato che è in corso di valutazione politica l'ulteriore prosecuzione del progetto di *project financing* relativo appunto ad un nuovo istituto e, nelle more, il Ministero della giustizia ha ultimato i lavori per le aule trattamentali ad uso dei detenuti. Lo stesso Ministero ha anche rappresentato che nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno in corso è stato inserito, per l'istituto di Bolzano, l'intervento di adeguamento delle sezioni detentive "ala sinistra" al DPR

Grazie, Ministro. Prendo atto del fatto che prendete sul serio la sensazione della nostra popolazione, che non si sente più sicura. Ogni tanto si sente dire: "sì, ma da voi, vicino ad Austria e Germania, è molto meglio che al Sud dell'Italia". Ma anche da noi ci sono tanti problemi, perché siamo una Provincia che è al confine, con tanti migranti senza permesso di soggiorno, che stazionano stazionano tutto il giorno in certe zone; la nostra popolazione quasi non ha più il coraggio di entrare in certi parchi o in certe zone della città. Pertanto, bene che lei abbia promesso di mettere più mezzi a disposizione, di rivedere la normativa quadro per la polizia locale e di fare in modo che il nostro carcere finalmente sia costruito.

Signor Ministro, ha destato scalpore nell'opinione pubblica quanto accaduto a Torino lo scorso 3 ottobre, quando, in occasione della partecipazione della Presidente del Consiglio alla giornata conclusiva del Festival delle Regioni e delle Province autonome, la polizia ha caricato il corteo composto da circa 250 persone, per la maggioranza maggioranza studenti, che la contestava pacificamente. Il corteo di studenti, partito da Palazzo nuovo, si è diretto verso Palazzo reale, prima di essere fermato dalle cariche della polizia. Numerosi video pubblicati *online* mostrano i manifestanti a volto scoperto e disarmati, fermi nel corteo innanzi al cordone di polizia, quando improvvisamente, fra le Forze dell'ordine, qualcuno dà l'ordine di caricare. I video mostrano le Forze dell'ordine colpire con i manganelli studenti giovanissimi del tutto inermi. Sono numerosi gli studenti, i manifestanti, i fotografi e i giornalisti che hanno riportato ferite durante gli scontri; diversi sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. Quanto accaduto è solo l'ultimo episodio di una serie, dopo oltre vent'anni dalla violenza del G8 di Genova. L'Italia non si è ancora dotata di una normativa che imponga i codici identificativi per le Forze dell'ordine, che avrebbe l'effetto di scoraggiare soprusi e identificare i colpevoli in caso di violazione delle norme, ma anche di isolare gli agenti violenti violenti tutelando l'operato della gran parte delle Forze dell'ordine che - ricordiamolo - agiscono nella legalità. Si consideri che nel 2012 l'Unione europea ha approvato una risoluzione che esortava gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo, come un *collar number* (numeri sul collo) o *shoulder number* (numeri sulla spalla): codici identificativi usati per riconoscere i singoli ufficiali di polizia, altrimenti impossibili da identificare in situazioni caotiche come gli scontri. Inoltre, nel 2016 è intervenuto anche il Consiglio sui diritti umani dell'ONU, che ha raccomandato che i funzionari delle Forze di polizia siano individualmente individualmente identificabili", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga ormai indifferibile l'introduzione nel sistema normativo di una disposizione che imponga l'adozione di codici identificativi e *bodycam* o comunque di strumenti atti all'identificazione degli agenti e a verificare le responsabilità individuali.

il costante contemperamento della tutela dell'ordine pubblico con l'esercizio delle libertà costituzionalmente garantite. Nel bilanciamento di tali esigenze, l'azione delle Forze di polizia privilegia sempre il dialogo e la negoziazione con i manifestanti, mentre l'uso della forza deve essere considerato un rimedio estremo per fronteggiare situazioni di particolare gravità caratterizzate da contesti di violenza o resistenza non altrimenti gestibili. Anche a Torino l'intervento delle Forze di polizia si è svolto in questa cornice ed ha consentito di garantire il regolare svolgimento di un evento pubblico con la presenza di autorità istituzionali e numerosi cittadini ai quali i manifestanti volevano impedire la partecipazione. Nello specifico, il servizio di ordine pubblico, nonostante le reiterate e violente provocazioni di alcuni noti agitatori che hanno cercato di strumentalizzare i giovani manifestanti, ha contenuto al minimo il rischio di incidenti. Segnalo a tal fine che, nei momenti di maggiore concitazione, oltre ad alcuni manifestanti che si sono fatti medicare sul posto, sono rimasti feriti quattro operatori di polizia. Con particolare riferimento alla questione del riconoscimento degli operatori di polizia, rappresento che nell'ordinanza di servizio che viene emanata dal questore per i servizi di ordine e sicurezza pubblica vengono indicati sia il funzionario di pubblica sicurezza responsabile della direzione del servizio che quelli addetti ai singoli settori di impiego. Aggiungo che, dal gennaio 2022, sono in uso al personale dei reparti inquadrati, impegnati nei servizi operativi, *bodycam* che costituiscono un utile strumento di documentazione degli accadimenti in occasione di eventi di rilievo che possono essere a rischio per l'ordine pubblico, e di identificazione anche degli agenti intervenuti. L'utilizzo di tali dispositivi è soggetto alle stringenti indicazioni relative ai dati sensibili, prescritte dal Garante della *privacy* al fine di tutelare i diritti delle persone oggetto delle riprese. Signor Presidente, signor Ministro, è inutile che dica che non ci riteniamo affatto soddisfatti della sua risposta; senza alcuna offesa, la riteniamo solamente fumo. È inutile che le ricordi che i video della manifestazione Da Torino sono pubblici e chiunque di noi può averli visti, quindi sappiamo che si trattava di una manifestazione non violenta e che i primi a caricare sono stati gli agenti. Signor Ministro, voglio semplicemente ricordarle che oggi, su ventisette sono già venti quelli che hanno adottato i codici identificativi e le *bodycam*; Nel nostro Paese le abbiamo, ma sappiamo benissimo che l'uso è a discrezione di chi comanda l'intervento e quindi delle volte non solo non servono a nulla, ma possono essere addirittura controproducenti. controproducenti. Infine, vogliamo ricordare che la nostra richiesta andrà avanti e che sarà a tutela non solamente delle possibili vittime di violenze e di soprusi, ma anche e soprattutto della stragrande maggioranza di uomini e donne che indossano una divisa e lo fanno con onore.

del nostro Gruppo e abbiamo ritenuto di doverla riproporre, perché gli episodi di cronaca hanno continuamente testimoniato che questa situazione, lungi dall'essere risolta, si è invece aggravata e quindi necessita di una risposta da parte del Governo.

una percezione che non può essere confutata semplicemente con dati matematici statistici, ma va presa in seria considerazione da parte del Governo. Quando il cittadino ha una percezione diffusa di pericolosità sociale, ciò ovviamente testimonia la necessità di un intervento. L'intervento del Governo nel perseguire gli autori degli illeciti

continuare a programmare interventi promozionali sul turismo, se poi non si dà la percezione, tanto ai cittadini quanto ai turisti, che le nostre stazioni ferroviarie, le nostre strade, le nostre città sono sicure.

a partire dal Forum delle Città metropolitane, da me costituito per un confronto costante su questi temi con i sindaci delle maggiori città, e dalla mia presenza in molteplici Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. In questa direzione si inquadrano, innanzitutto, le operazioni cosiddette ad alto impatto, che rafforzano la nostra capacità di controllo dei luoghi pubblici a elevata concentrazione di persone, riducendo l'insicurezza percepita e aumentando l'efficacia dell'azione repressiva. Dall'inizio dell'anno, nell'ambito di questa modalità di controllo del territorio e di prevenzione generale, che costituisce ormai un dispositivo consolidato e sistematico, sono stati effettuati 677 interventi, di cui 307 presso stazioni e aree limitrofe. Sono state impiegate circa 41.500 unità delle Forze di polizia, col supporto di ulteriori 5.000 unità di polizia locale, di personale delle aziende sanitarie locali, delle aziende municipalizzate e dell'ispettorato del lavoro. Sono state controllate oltre 384.000 persone, di cui 809 arrestate e 4.771 denunziate. Sono stati inoltre adottati 933 provvedimenti di espulsione nei confronti di stranieri, controllati più di 47.000 veicoli e oltre 87.000 esercizi pubblici. Aggiungo, peraltro, che il recente decreto-legge n. 133 del 2023 ha previsto il rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi dove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, attraverso l'incremento di ulteriori 400 unità dedicate a tale specifico impiego nell'ambito del contingente delle Forze armate per l'operazione Strade sicure. Per avere un quadro aggiornato delle criticità e delle esigenze, dopo i fatti di Caivano, ho inviato ai prefetti una direttiva per la mappatura delle aree più gravemente degradate e più bisognose di analoghi interventi. Sono consapevole che il lavoro delle Forze di polizia è fondamentale e che, però, non basta. Occorre agire per rimuovere le cause del degrado e della crescente emarginazione sociale, che alimentano fenomeni di illegalità e insicurezza. Pertanto, ritengo essenziale la costante interlocuzione e collaborazione con i sindaci, che vanno sostenuti anche sul versante delle loro specifiche attribuzioni in materia di servizi sociali e interventi di riqualificazione urbana. Informo, infatti, che per Roma, Milano e Napoli abbiamo messo in campo una specifica contribuzione, a valere su fondi del Ministero dell'interno, per sostenere le amministrazioni comunali nelle iniziative dirette a contrastare gravi forme di marginalità sociale. È questa la direzione che ho voluto imprimere al rapporto con i primi cittadini, verso la quale stiamo orientando anche la destinazione di importanti risorse, attingendo in particolare al fondo per la sicurezza urbana, con l'obiettivo di conseguire risultati concreti positivi e duraturi. Questa strategia, la strategia del Governo, si sta muovendo su più piani, con azioni di breve, medio e lungo periodo, che affiancano alle operazioni di contrasto, destinato a proseguire in modo sistematico, iniziative sul piano economico, sociale, educativo e culturale volte a riqualificare le nostre città e ad affermare pienamente legalità e sicurezza. Signor Ministro, voglio innanzi tutto darle atto di lavorare nella direzione di un rafforzamento sul tema della sicurezza delle nostre stazioni e, più in generale, delle città. Non è il suo impegno a essere in discussione. È anche vero, però, che la situazione è particolarmente complessa e, quindi, nessuno vuole fare demagogia. Penso però che la sicurezza, contrariamente a certa a sinistra, sia un valore per tutti,

Le devo dire che, nonostante la sua risposta fosse già stata data al nostro Gruppo in passato, noi questa percezione di un miglioramento non la vediamo e le faccio un esempio molto chiaro davanti a tutti: Roma Roma è in una situazione in cui, quando si arriva alla stazione, non si ha la sensazione di essere in sicurezza e dove il tema del degrado è davanti a tutti per una serie di fattori, ivi compreso il fatto che vi è ormai una costante coda in

o qualsiasi altra città d'Italia è di misurare i dati che ha riportato sulla reale efficacia delle azioni che si stanno intraprendendo, considerando certamente che a questo va sempre accompagnato

una mera elencazione di dati che sembrano andare verso una direzione di miglioramento in realtà non corrisponda alla reale

*(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, i dati relativi al primo semestre del 2023 della banca dati interforze del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ci dicono

Innanzi tutto, i reati che variano vedono le città di Milano, Venezia e Roma capeggiare le classifiche per il furto con destrezza; i furti in abitazione vedono in cima alla classifica la città di Pisa (con 420 casi su 100.000 abitanti), la città di Pavia (con 390 casi casi su 100.000 abitanti) e invece ci sono pochi furti in abitazione nella provincia di Oristano (con 60 casi ogni 100.000 abitanti). Poi arriviamo ai furti delle autovetture: in questo caso la classifica vede primeggiare la Provincia di Barletta-Andria-Trani con 1.036 casi su 100.000 abitanti; la Provincia di Foggia a seguire con 638 casi e poi la Provincia di Napoli. I furti di auto, invece, sono limitati nelle Province di Sondrio, Belluno e Pordenone.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, per esempio, una delle ultime Province nate, la cui questura è stata istituita nel luglio del 2021 come anche tutti i comandi provinciali, sconta oggi una presenza sottodimensionata di personale delle forze pubbliche, come viene anche evidenziato dall'analisi criminale redatta dal circondario della procura della Repubblica di Trani proprio di recente, nel settembre del 2023. Come anche sono sottodimensionate le questure delle Province di Roma, Rimini e Milano. Si chiede, signor Ministro, di sapere quali siano le valutazioni in merito a questa differenziazione e alle diverse emergenze esistenti sul territorio e quali siano le soluzioni che il Ministro intende adottare prossimamente, soprattutto per cercare di tutelare i nostri cittadini e per dare delle risposte a queste ultime

Signor Presidente, il dato aggregato sulla delittuosità a livello nazionale indica che nei primi otto mesi del 2023 si registra una lieve flessione, - 0,4 per cento, rispetto all'analogo periodo del 2022, ma più che la statistica, come lei ha detto, conta l'approccio generale al problema della sicurezza. In questo senso evidenzio che l'Italia, com'è stato detto, ha territori con caratteristiche ed esigenze assai diverse. A tali peculiarità una buona politica deve prestare attenzione nell'elaborazione delle proprie strategie a partire proprio dalle politiche di sicurezza. Servono dispositivi flessibili e commisurati ai contesti e ai bisogni dei territori e una metodologia di intervento basata su logiche di rete. È proprio in segno di attenzione alle specificità dei territori che ho deciso di presiedere - ne ho fatti già tanti personalmente - in alcune realtà connotate da particolari criticità, i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. presieduto tali riunioni in diverse città del Paese. Ancora ieri sono stato a Cagliari e ho ancora intenzione di recarmi in altre città. A breve andrò proprio a Barletta, città da lei citata, senatore. Sono infatti convinto che una strategia di sicurezza integrata richieda una costruttiva e leale collaborazione con gli amministratori locali e la linea di azione del Governo mira proprio ad armonizzare esigenze diverse e tutte meritevoli di attenzione, perché da un lato bisogna combattere l'illegalità e restituire sicurezza ai cittadini, dall'altro occorre puntare su una rigenerazione e riqualificazione urbana come volano di uno sviluppo equo e sostenibile. Inoltre, credo vada sottolineato che l'attenzione del Governo non si rivolge unicamente alle aree metropolitane ma tiene sempre conto e valorizza i bisogni e la domanda di sicurezza dei centri urbani minori, anche grazie alla sistematica azione di coordinamento delle Forze di polizia svolta a livello locale dalla rete dei prefetti. Sul piano degli strumenti ritengo non si possa prescindere da un adeguato potenziamento delle risorse umane strumentali delle Forze di polizia. Con la prima legge di bilancio di questo Governo - l'ho detto anche prima in un'altra risposta - sono già state assunte importanti iniziative in questa direzione ed altre ne prenderemo. Per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza sono state previste, a legislazione vigente, complessivamente nei rispettivi piani pluriennali di assunzione straordinaria, 18.148 unità da assumere. Sono stati già assunti 11.503 operatori e, nel corso dei prossimi anni, sarà possibile immettere in servizio altre 6.645 unità di personale. Quindi abbiamo intenzione di continuare continuare lungo questa strada assicurando il necessario sostegno alle Forze di polizia, nella ferma convinzione che si tratta di un investimento in legalità, sviluppo e democrazia. Il nostro impegno ad incrementare le risorse proseguirà anche nella prossima legge di bilancio, come dicevo, anche in vista dei grandi eventi che il nostro Paese dovrà organizzare. Oltre a ciò, proseguiremo l'esperienza assai positiva delle operazioni ad alto impatto, di cui pure ho parlato prima, e siamo impegnati a contrastare l'illegalità in ogni sua manifestazione, da quella delle occupazioni abusive degli immobili e della criminalità predatoria, fino alle più gravi pratiche delittuose della criminalità organizzata. Tutto questo perché il Governo ha ben chiaro che la sicurezza è un bene primario per il futuro del Paese e intende garantirlo pienamente. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Damiani,

- Premesso che sabato 7 ottobre 2023 l'organizzazione terroristica palestinese Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha dato inizio ad un violentissimo attacco via mare, via terra e via aria nei confronti di Israele, che ha provocato oltre mille morti tra la popolazione israeliana; dalle ultime notizie di stampa, si apprendono deplorevoli crimini ai danni di civili israeliani, che riportano alla mente le immagini dei più violenti attacchi terroristici subiti dalla popolazione europea nel corso degli ultimi decenni; considerato che: l'attacco rischia di ridare vigore alla minaccia jihadista globale; tale potenziale minaccia rende necessario l'innalzamento del livello di attenzione verso ogni possibile obiettivo e un rafforzamento delle misure di prevenzione sul territorio; la nuova ondata di violenza nei confronti di Israele non può essere circoscritta ad una dimensione locale, ma va considerata in un quadro di instabilità internazionale che rischia di acuire nuovamente lo scontro confessionale in Medio Oriente, e conseguentemente la mobilitazione delle organizzazioni fondamentaliste; il proliferare delle manifestazioni, dal carattere ambiguo, osservate nelle principali città europee, nella cornice di un generico sostegno alla causa palestinese, ha evidenziato altresì l'acuirsi di un sentimento d'odio nei confronti di Israele mai sopito negli anni; come si apprende da organi di stampa, è all'attenzione del Governo italiano un piano di sicurezza antiterrorismo; si ritiene necessario che all'interno del piano siano previste azioni di contrasto all'immigrazione clandestina, vista come potenziale veicolo del fondamentalismo islamico, in accordo con l'Unione europea e con le principali organizzazioni multilaterali internazionali, si chiede chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo stia adottando in relazione a quanto illustrato. PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Signor Presidente, a seguito dell'attacco subito da Israele già nella giornata di sabato scorso, è stato immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale e nella seduta del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ho convocato d'urgenza lo scorso 10 ottobre, alla quale hanno partecipato anche le agenzie di sicurezza, sono state approfondite le possibili minacce e gli strumenti di prevenzione e contrasto. All'esito dell'incontro è stato ulteriormente innalzato il livello di attenzione e rafforzate le misure di prevenzione generale, con particolare riguardo alle aree di maggior transito e all'adozione di misure di difesa passiva dei siti sensibili. In attuazione degli indirizzi impartiti, le prefetture hanno già disposto l'intensificazione delle misure a protezione degli obiettivi sensibili e dei dispositivi di prevenzione sul territorio. La minaccia terroristica, inoltre, è alla costante attenzione del Comitato analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, che si è riunito appositamente, anch'esso dal 10 ottobre, per valutare l'evoluzione dei profili di rischio anche nei contesti antagonisti e nell'ambiente penitenziario. Aggiungo che l'azione del Governo, sin dal suo insediamento, si è incentrata su ogni forma di contrasto all'immigrazione irregolare, anche in relazione ai possibili profili di rischio di infiltrazione terroristica nei flussi. I recenti tragici avvenimenti impongono una rinnovata e più elevata attenzione, senz'altro, in particolare attraverso il potenziamento delle attività interforze per i controlli delle frontiere e di quelle effettuate dalle specifiche *task force* operanti nelle principali aree di sbarco e negli *hotspot* nazionali. In questo senso ho dato specifiche direttive - quindi la rassicuro in tal senso - per l'intensificazione di ogni raccordo informativo tra le Forze di polizia e le agenzie di *intelligence*, al fine di monitorare l'evoluzione del conflitto e i suoi possibili riflessi sui flussi migratori, sugli ingressi e sulle presenze nel territorio nazionale.

Come premesso nel quesito, è evidente che, se la questione sbarchi e flussi migratori assumerà anche un carattere securitario, si rende necessario un coinvolgimento delle principali istituzioni internazionali nell'arginare tale fenomeno, a tutela della sicurezza dell'intero continente europeo. Inoltre, il secondo concetto che vorremmo esprimere riguarda l'ambiguità di alcune comunità islamiche presenti in Europa, ma non solo. Abbiamo visto immagini di manifestazioni da New York a Sydney, passando per le principali città europee, con slogan, canti e insulti contro Israele, la sua legittimità e contro il popolo ebraico. L'*escalation* del conflitto israelo-palestinese può contribuire ad alimentare le varie spaccature in Medio Oriente e a cascata fomentare alcune organizzazioni islamiste in grado di operare a livello globale. Anche per tale ragione ribadiamo l'urgenza di sostenere processi diplomatici in grado di congelare il conflitto nel breve. Ma soprattutto ribadiamo il sostegno alle iniziative in grado di portare i principali Paesi arabi ad una normalizzazione con Israele. Un ambiente cooperativo e non conflittuale in Medio Oriente rimane la principale garanzia per impedire le esplosioni di focolai di instabilità che - come la storia ci insegna - comportano la moltiplicazione della minaccia del terrorismo globale. Siamo lieti di sapere, tramite le sue parole, che il Governo, a fronte dello scoppio di una nuova crisi, si è prontamente impegnato per gestire le potenziali minacce. La ringrazio nuovamente per la risposta e le auguriamo buon lavoro.

*(PD-IDP)*. Signor Ministro, i fatti sono noti, o perlomeno una parte degli stessi. A seguito di un decreto-legge di questo Governo, il cosiddetto decreto Cutro, che sin dall'inizio, anche sotto il profilo giuridico, ha presentato falle e criticità, sono arrivate - come era prevedibile e previsto - le prime pronunce delle preposte autorità giudiziarie, che non hanno convalidato i provvedimenti di trattenimento. Signor Ministro, oggi noi non parleremo sul merito dei provvedimenti dei giudici, sui quali lei ha dichiarato che legittimamente proporrà impugnazione e dei quali deve leggere ancora le motivazioni, anche se la sua compagine di Governo, a principiare dalla Presidente del Consiglio, nell'immediatezza dei fatti si è scandalizzata che la giurisdizione disattendesse con i suoi provvedimenti la linea politica e programmatica di questo Governo. Vorremmo invece parlare del fatto che successivamente un Ministro di questa Repubblica, il ministro Salvini, ha pubblicato un video dove era inquadrata una magistrata presente a una manifestazione pubblica di ben cinque anni fa. Ha utilizzato questo video per attaccare la singola magistrata, chiedendone le dimissioni e finanche sanzioni disciplinari. Pertanto, noi oggi non parleremo dell'opportunità di presenziare da parte di magistrati a manifestazioni pubbliche, sebbene secondo la Costituzione non può essere preclusa ad alcun cittadino la possibilità di esprimere opinioni e pensieri, perché l'indipendenza e la terzietà dei medesimi va valutata sulla base dei provvedimenti che vengono assunti e delle motivazioni poste alla base dei provvedimenti - solo dei provvedimenti - giammai facendo uno *screening* del passato della vita di un magistrato. Se è condivisibile l'affermazione secondo la quale ogni magistrato deve essere comunque sempre percepito come figura al di sopra dello scontro politico-partitico, tuttavia non possiamo non rilevare e sottolineare quanto segue. Indipendentemente da qualunque valutazione sull'opportunità di presenziare a manifestazioni pubbliche, tale partecipazione non deve e non può comunque in alcun modo motivare o giustificare aggressione personali, delegittimazioni di singoli magistrati della magistratura. Lo ha detto anche Giovanni Maria Flick, già Ministro della giustizia e giudice emerito della Corte costituzionale. Giudicare una sentenza dalla vita del magistrato e non dai suoi argomenti ci porta fuori dalla civiltà giuridica e, dunque, oggi il punto è ancora soltanto il seguente: la manifestazione si è svolta nel 2018, cinque anni fa. Ancora oggi rimane da chiarire come sia stato conservato e soprattutto diffuso il video. Non ci hanno per niente rassicurato le dichiarazioni del sottosegretario sottosegretario Molteni ieri, che ha dichiarato che non esistono video ufficiali, che c'è un carabiniere che si era indicato come autore del video, ma che ha ritrattato; e poi le agenzie di stampa ci hanno detto che il carabiniere ha negato di aver mai confessato di essere l'autore del video. video. Oggi vogliamo sapere da lei, signor Ministro, senza reticenze e senza omissioni, se non ritenga necessario e urgente intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di chiarire la precisa ricostruzione dei fatti, le modalità con le quali i filmati sono stati registrati, acquisiti, entrati

siano accessibili, al fine di garantire che non sia in alcun modo violato il pieno godimento da parte di tutti i cittadini di tutte le garanzie costituzionali.

che il video in questione che ritrae il giudice Iolanda Apostolico nella manifestazione pubblica al porto di Catania il 25 agosto del 2018 non proviene da documentazione della questura di Catania. In In alcuno degli atti redatti all'epoca dal personale impiegato nei servizi di ordine pubblico e a seguito dei fatti verificatisi nel corso della manifestazione è menzionata la dottoressa Apostolico. La questura di Catania, a seguito di quella manifestazione pubblica, dopo aver acquisito le riprese video effettuate dalla Polizia scientifica, inoltrò il 21 settembre di quell'anno una segnalazione all'autorità giudiziaria, senza individuare responsabilità penale da parte dei partecipanti alla manifestazione. È notorio, ed è stato più volte precisato, che i fatti attinenti alla recente diffusione di video riguardanti la manifestazione in questione sono ora all'attenzione della procura della Repubblica di Catania. Le modalità di raccolta, conservazione e trattamento dei dati acquisiti dalle forze di Polizia nei servizi di ordine pubblico sono disciplinati dal regolamento n. 15 del 2018 e dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 e sono consentiti dal regolamento appena citato per documentare specifiche attività preventive o repressive di reati, nonché situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica, laddove ritenuto poi necessario. Evidenzio ancora una volta che, sulla base di tale quadro normativo, gli uffici di Polizia non detengono, né tantomeno conservano video o immagini non ufficiali e che, per quanto riguarda le riprese non utili effettuate durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica, non esiste un archivio informatico o una banca dati per la loro conservazione. Sottolineo infine che le immagini video raccolte dalla Polizia di Stato non sono sottoposte a elaborazioni informatiche a fini identificativi. Che dire, Ministro? Dopo le sue parole rimane - per usare un lessico caro dalle parti del Viminale - un carico residuale di opacità, silenzi e oscurità. Chi ha girato quel video? Come l'ha avuto il ministro Salvini? Com'è possibile che, dopo cinque anni, subito dopo la sentenza, spunti un video mirato e si scateni una manganellatura mediatica contro una magistrata? Abbiamo detto anche noi - Anna Rossomando lo ha ripetuto - che è meglio se un magistrato, pur avendo diritto - e ci mancherebbe - di esprimere le opinioni e vivere il suo tempo e la società, non partecipi a manifestazioni. "Può ma non deve", ha detto il Ministro: su questa frase potremmo trovare un accordo. La terzietà deve esserci e deve essere anche percepita. Ma detto questo, è a quelle domande che sono state poste che in un Paese democratico si devono dare risposte. Voi non le date, ma del resto membri del Governo come un Sottosegretario alla giustizia hanno già usato carte riservate per colpire e diffamare le opposizioni. Si chiama squadrismo, ma qui c'è qualcosa di ancora di più grave.

un clima intimidatorio e - attenzione - questo vale per tutti. Un magistrato deve agire con serenità, pur avendo le proprie intime convinzioni. Ma sulle sentenze, senza - è stato detto avere né timori di ripercussioni sulla sua carriera, né speranze di promozione: deve solo agire secondo la legge. Per questo siamo profondamente insoddisfatti. Non prendetevela con i magistrati che fanno sentenze, non solo a Catania. Prendetevela con voi stessi, con la vostra fallimentare politica sui migranti, con le vostre leggi e i vostri decreti, che violano norme e direttive europee e violano i principi di umanità.

Signor Ministro, sono passati cinque mesi da quando la Romagna è stata colpita da una delle peggiori alluvioni degli ultimi anni; oltre 5 miliardi di metri cubi d'acqua sono venuti giù in quei giorni terribili di maggio. Risuonano ancora le promesse della presidente Giorgia Meloni: "Risarciremo al 100 per cento chi è stato danneggiato". Sono parole che, almeno ad oggi, suonano come una beffa per tutti quei cittadini e quelle imprese che hanno preso pochi spicci o niente. Sono molti i temi su cui il Governo dovrebbe dare spiegazioni ai romagnoli colpiti dall'alluvione di maggio e chiedere scusa per l'incapacità e l'inadeguatezza, a partire dagli inaccettabili ritardi fino alle insufficienti risorse stanziate per la ricostruzione. Questa interrogazione pone l'attenzione su un tema preciso, che incontra il nostro futuro: quello delle scuole. È proprio perché si parla di bambini e di giovani che le mancanze e le bugie sono ancora più intollerabili e inaccettabili. A seguito dei gravissimi episodi di violenza avvenuti a Caivano, sono state introdotte norme finalizzate a risanare e a riqualificare un territorio in un contesto urbano particolarmente disagiato. Sono previsti interventi volti a rafforzare l'offerta educativa nelle scuole del Meridione, caratterizzate da dispersione scolastica. In tal senso, le scuole di tali Regioni possono attivare contratti per personale ATA fino al 31 dicembre 2023 e non fino alla fine dell'anno scolastico. La relazione tecnica sostiene letteralmente che per gli stessi non sono previste proroghe. Le risorse per il personale ATA aggiuntivo non costituiscono peraltro nuovi stanziamenti e quei 10 milioni di euro provengono dai fondi destinati alle scuole dei territori colpiti dall'emergenza dell'Emilia Romagna. Lì ci sono tantissime scuole che sono ancora molto in difficoltà. Il suo Ministero specifica che trattasi di economie, in quanto gli interventi per le scuole dei territori alluvionati erano ammissibili entro la data del 31 agosto. Ma il decreto-legge n. 61 del 2023, all'articolo 5, comma 1, prevede l'istituzione prevede l'istituzione del fondo predetto per tutto l'anno 2023. Il riparto delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche dei territori coinvolti nell'emergenza avrebbe dovuto essere stabilito con un decreto che concerne il suo Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ebbene, quel decreto non è stato adottato entro agosto, ma solo dopo lo scoppio di questa polemica. Insomma, nonostante lo stanziamento fosse dedicato per l'anno 2023, con il decreto-legge Caivano i fondi sono stati utilizzati per altre finalità. Le chiedo, Ministro, se è a conoscenza di questa situazione e quali sono le misure che intende intraprendere il Ministero per garantire il ripristino delle risorse sottratte dai fondi dedicati alle scuole dell'Emilia Romagna e per assicurare, dall'altra parte, un piano

qui oggi. In legge di bilancio troverà su questo posizioni specifiche da parte del MoVimento 5 Stelle. Signor Presidente, gentili senatori, con riferimento al riparto dei fondi stanziati a favore delle scuole dell'Emilia Romagna coinvolte negli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, intendo chiarire subito che tutte le scuole interessate hanno ricevuto in tempi brevissimi esattamente quanto da loro richiesto. Ricordo, infatti, che con il decreto-legge n. 61 del 2023 è stato istituito un fondo speciale, della consistenza di 20 milioni di euro, rivolto a consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica regolare attività didattica (attività che è tempestivamente ripresa). Con tali risorse, dunque, erano ammissibili interventi, entro la data del 31 agosto, finalizzati alla sola fase della prima emergenza. Abbiamo previsto, per agevolare e velocizzare gli interventi delle scuole, importanti semplificazioni procedurali. Ai fini del riparto del predetto fondo, il Ministero ha ritenuto doveroso acquisire immediatamente il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche interessate, che hanno formulato richieste per un importo complessivo pari a 10,174 milioni: sostanzialmente le scuole hanno chiesto 10,174 milioni di euro rispetto ai 20 stanziati. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi, il Ministero ha avviato una procedura eccezionale straordinaria volta ad ottenere un'anticipazione di tesoreria da Bankitalia, che ha consentito già dal 20 giugno 2023, dunque a soli venti giorni dall'adozione del decreto-legge, di erogare le risorse finanziarie alle scuole nelle more del decreto di riparto, la cui adozione, peraltro imminente, rappresenta un adempimento formale dal momento che l'attribuzione sostanziale delle risorse è già avvenuta. Aggiungo che, decorso il termine del 31 agosto 2023, quindi soddisfatto integralmente il fabbisogno espresso dalle scuole interessate dall'alluvione, la parte del fondo non utilizzata, pari ad euro 9,825 ha rappresentato un'economia che, qualora non impiegata entro l'anno, non sarebbe stata più utilizzabile. Ricordo infatti che, come dovrebbe sapere chiunque conosca le nozioni di base della contabilità pubblica, la stessa natura di queste risorse, in quanto spese di parte corrente, non avrebbe in alcun modo consentito un reimpiego oltre l'anno 2023 in interventi di investimento quali sono quelli per l'edilizia scolastica (parte corrente e investimento su due cose molto diverse). Per tale motivo ho ritenuto opportuno impiegare tali economie, che altrimenti sarebbero state perse, per finanziare il potenziamento dell'organico del personale ATA disposto con il decreto Caivano (decreto-legge n. 123 del 2023). A tal riguardo, in merito alla scadenza dei contratti per detto personale, intendo chiarire che il termine fissato al 31 dicembre 2023 risponde ad una ragione contabile - ancora una volta una ragione contabile - dovuta al fatto che le risorse utilizzate in quanto residui di fondi del Ministero sono collegate a questo anno solare e solo a questo anno solare. Ciò, beninteso, in attesa delle misure di natura pluriennale che potranno essere disposte solo con legge di bilancio. Signor Ministro, devo dire che la sua risposta purtroppo non mi soddisfa e devo in parte smentirla, perché comunque le risorse di cui stiamo parlando erano destinate all'Emilia-Romagna e potevano essere spese entro il 31 dicembre *(Applausi)*, quindi le scuole potevano ancora fare accesso a quei fondi se voi non li aveste distolti e spostati su un altro capitolo. Capisco che non sapete come fare e dove reperire le risorse - ce l'avete già detto - in tantissimi campi, ma non è una scusante per eliminare soldi da un territorio bisognoso e girarli a un altro altrettanto bisognoso. La data del 31 agosto era per la spesa in deroga rispetto alle norme sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni, ma c'erano istituzioni che potevano seguire i percorsi normali non in deroga e farlo entro la fine dell'anno; voi avete tolto questa possibilità spostando i soldi dalle scuole colpite dall'alluvione a un altro capitolo di spesa. Purtroppo conosciamo bene questo vostro *modus operandi*. Sbandierate le risorse per il mondo della scuola, ma sono fondi esistenti che spostate da un'altra parte. Avete erogato solamente 200 milioni di risorse vere anzi, meno di 200 milioni - nel 2023 per l'istituzione scolastica: nulla a confronto dei 10 miliardi che aveva erogato il Governo Conte II in un solo anno per rispondere alle emergenze della scuola; nulla rispetto ad altri investimenti. La media europea della spesa rispetto al PIL sull'istruzione ma noi siamo ben lontani da questo livello di spesa. Perché, signor Ministro, non si impegna a portare i nostri investimenti al pari della media europea? Perché non si impegna, innanzitutto, a trovare le risorse per prorogare i contratti ATA fino alla fine dell'anno scolastico? Sappiamo bene che la contabilità ragiona per anni solari. Ma il Ministero il Ministero dell'istruzione ha delle risorse pluriennali, proprio perché lavora su anni scolastici, che vanno a cavallo di due anni. Quindi, siete voi che, ancora una volta, siete incapaci di trovare le risorse per l'istruzione. *(Applausi)*. Parlate di lotta alla dispersione, ma state ridimensionando la rete scolastica, tagliando nell'ambito delle autonomie e il numero dei dirigenti scolastici. Scaricate il peso dei tagli sui territori, già in difficoltà e fragili. Soprattutto, non c'è alcun intervento educativo vero. Non c'è coinvolgimento di famiglie e del terzo settore. Con il Governo Conte avevamo istituito i patti educativi di comunità, una leva generativa per i territori, un'alleanza di comunità tra scuole, famiglie e terzo settore. Abbiamo presentato una proposta di legge al riguardo. La prego di leggerla, signor Ministro. La scuola ha bisogno di un approccio diverso da quello muscolare che vi ha contraddistinto fino ad oggi. Le sanzioni, da sole, sono una bandierina piantata nel deserto.

oggi è il 12 ottobre, una data importantissima per la storia del mondo occidentale: il 12 ottobre 1492 fu scoperta l'America.

con sé le radici greco-romane della nostra cultura, noi abbiamo costruito quell'asse che poi ha congiunto l'Europa con l'America, creando quel mondo occidentale che, a volte, ci sembra quasi in pericolo e che ci sembra noi dovremmo difendere. dovremmo difendere. Noi non dobbiamo rimanere inerti dinanzi alla *cancel culture*, che tende a far sì che i nostri bambini dedichino magari tutta la terza elementare allo studio dei famigerati dinosauri; in quarta elementare abbiano un'infarinatura su fenici e babilonesi; in quinta velocemente e fugacemente studino l'antica Roma, per poi andare avanti alle medie. Sarebbe utile, signor Ministro, che si ritornasse all'era precedente alle riforme che si sono susseguite in quest'ultimo decennio decennio e si restituisca ai nostri bambini la possibilità di sedimentare, di conoscere entro la quinta elementare la periodizzazione della storia; che gli si consenta di conoscere quelli che sono gli eventi storici fondamentali; che gli si restituisca la conoscenza di quelle radici

va anche a ledere e a indebolire l'identità e la conoscenza profonda che il nostro popolo ha e che deve continuare ad avere.

oggetto di insegnamento nelle scuole, che prima si definivano programmi, è stata sostituita da tempo da un modello incentrato sugli obiettivi formativi e sui traguardi di competenza attesi per ogni grado di istruzione. la periodizzazione unica dei contenuti e delle tematiche afferente alla storia e alla geografia per ogni ciclo di istruzione, introdotta con le indicazioni per il curricolo del 2007, è stata confermata, da ultimo, dalle indicazioni nazionali del primo ciclo del 2012. La modifica della progressione dei contenuti, degli obiettivi e dei traguardi per le discipline di storia e geografia sarà dunque valutata nell'ambito della revisione delle predette indicazioni nazionali, la cui definizione richiede, ovviamente, il necessario coinvolgimento della comunità scolastica. Al riguardo, intendo chiarire che per me la scuola deve sviluppare nelle studentesse e negli studenti un pensiero critico con cui affrontare la complessità del nostro tempo in un mondo in continuo cambiamento. A tale scopo, risulta centrale lo studio della storia e della geografia, che fornisce gli strumenti cognitivi necessari per capire da dove veniamo, chi siamo e dove vogliamo andare. Non vi è dubbio infatti che, per comprendere e definire il ruolo che intendiamo ricoprire, sia come individui, sia come comunità, sia indispensabile approfondire lo studio delle culture dei periodi che hanno maggiormente caratterizzato la nostra civiltà, come pure conoscere società, economie, istituzioni e cultura dei Paesi moderni.

non sia assicurato appieno nell'intero ambito della scuola dell'obbligo. Tanto premesso, intendo rassicurare sul fatto che la questione è all'attenzione del Ministero, che ha costituito un gruppo di lavoro sulle discipline umanistiche volto proprio ad approfondire quelle istanze di rinnovamento nella didattica di dette materie, la cui rilevanza è testimoniata tra l'altro dalla stessa attenzione rivolta dai senatori interroganti in questa specifica occasione. Signor Ministro, ho ascoltato con interesse questa sua risposta e sono certa, quindi, che riusciremo ad ottenere questa riforma così attesa e rilevante. Pensi che mio fratello, che è un professore universitario nel Regno Unito, non perde mai occasione di ricordarmi quanto all'estero

le radici in profondità, ma che devono essere da noi potate e innaffiate per farne un domani alberi forti, potrà portare nuovamente ad avere una popolazione con una identità, una consapevolezza e una conoscenza forti delle proprie radici e quindi ben orientata per il futuro.

ci ha lasciato don Josef Hurton, all'età di novantacinque anni. Si può ben dire che sia stato in Alto Adige e in Italia l'ideatore del soccorso alpino e l'inventore dei cani da valanga. Nacque nel 1928 a Bratislava, nell'odierna Slovacchia. Frequentò le scuole elementari in Austria, le medie in Ungheria e il ginnasio-liceo in Cecoslovacchia, dove nel 1949 fu internato in un campo di lavoro, da cui riuscì a fuggire nel 1950. Trovò protezione nella chiesa, presso il nunzio apostolico a Vienna. Completò gli studi alla Pontificia Università Lateranense di Roma per studiare poi scienze orientali all'Università Gregoriana sempre di Roma, lingue e letterature straniere a Padova e arte orientale a Bologna. Nel 1955 venne ordinato sacerdote e venne mandato in Alto Adige, dove lavorò dal 1956, prima a San Leonardo in Badia, poi a Sesto. Il 2 agosto 1960 fu mandato a Solda, a sostituire il parroco rimasto sotto una slavina e il cui corpo venne recuperato tre mesi e mezzo dopo, grazie al fiuto di un cane. Proprio quella tragedia ispirò anche la sua scelta di vita, quasi una seconda vocazione: l'impegno nel soccorso alpino, che allora non esisteva. Fu parroco di Solda fino al 1999 e vi rimase per il resto della sua vita; fondò la scuola per cani da valanga di Solda, guidandoli anche personalmente. Promosse il servizio di elisoccorso, appoggiandosi e coinvolgendo il comando delle truppe alpine con i mezzi militari. Fu anche regista e autore di libri, girava e proiettava film in sedici millimetri e li mostrava agli ospiti e alle gente del posto, durante serate cinematografiche da lui stesso organizzate. Nella sua vita ha recuperato oltre 200 vittime di incidenti mortali in montagna. Davanti a ogni cadavere recitava una preghiera, perché quello era non un pezzo di legno, ma un essere umano che avrebbe Don Hurton si fermava volentieri a dialogare sulla bellezza del creato e sull'importanza del rispetto per la montagna con i tanti villeggianti attirati dalla catena dell'Ortles. Diceva: gli ospiti arrivano da noi stressati e vogliono ricrearsi sia fisicamente che spiritualmente. Noi dobbiamo cercare di supportarli, prendendoli per come sono e facendo di tutto perché possano tornare a casa migliori e rigenerati. Il suo modello di carità si esprimeva poi nel primo annuncio ai familiari delle vittime in montagna: meno parole si usano meglio è. Quando si verificano tragedie gravi, magari mortali, noi dobbiamo essere soprattutto presenti e partecipi, affermava. Ora la sua terra lo ricorda con il rispetto che è riservato a chi ha lasciato doni eterni. L'Ortles e il Gran Zebrù sono state le sue amate montagne e continueranno a vegliare su di lui. *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'epoca storica, nelle more dell'emergenza da Covid-19, i nostri giovani vivono un momento di disagio e sono costantemente bombardati da stimoli esterni e sottoposti a pressioni pressioni sociali. Tutto ciò crea un senso di incertezza riguardo al loro futuro. Pertanto viviamo in un'epoca in cui le sfide psicologiche sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, dei grandi e dei piccoli. In questo contesto si rende necessario introdurre l'educazione emotiva come strumento essenziale per aiutare gli studenti a comprendersi, a comprendere i propri compagni e ad affrontare la complessità della vita. Badate bene: non sto facendo discorsi utopistici, perché negli altri Paesi europei ciò che sto dicendo è già realtà: dalla Finlandia ai Paesi Bassi, dall'Inghilterra alla Svezia, moltissimi Stati membri già hanno integrato l'educazione emotiva nel proprio sistema educativo e molti altri stanno seguendo il loro esempio. Onorevoli colleghi, immaginate un mondo in cui ogni giovane ha una consapevolezza profonda di sé stesso e degli altri, in cui si sente capito e capace di capire, in cui le emozioni non sono viste come una debolezza da nascondere, ma come una forza da coltivare. Questo è il mondo che possiamo creare attraverso l'introduzione dell'educazione emotiva nelle scuole. Ebbene, quando insegniamo ai nostri giovani ad affrontare le sfide emotive stiamo costruendo le basi per una società più compassionevole, non indifferente e rispettosa dell'altro, perché l'empatia e la comprensione reciproca devono ritornare ad essere elementi centrali nel nostro villaggio globale. Molti ricorderanno il libro «Villaggio Globale» di Mcluhan. Un cittadino che si prende cura del prossimo, dei più deboli, di tutti gli esseri viventi e di tutta la natura, quella natura che è parte integrante della vita dell'uomo e che costituisce l'ossatura su cui si fonda l'esistenza stessa. Per realizzare questa visione dobbiamo agire insieme come comunità, genitori e insegnanti, amministrazioni scolastiche e soprattutto noi istituzioni, perché l'educazione emotiva diventi una priorità nelle nostre scuole. Onorevoli colleghi, siamo chiamati a essere i custodi del futuro di milioni di studenti, che saranno gli uomini del domani, cioè siamo chiamati a creare un mondo in cui le emozioni siano considerate una risorsa preziosa. Perciò non come senatrice, ma da ex insegnante, da madre, da cittadina chiedo a questa maggioranza di introdurre l'educazione emotiva nelle scuole, aumentando il monte ore almeno di un'ora a settimana e lasciare un'eredità di comprensione con passione e benessere per le generazioni future. Soprattutto in questo momento storico in cui la guerra viene considerata come strumento per definire gli assetti geopolitici, abbiamo il dovere civico e morale di riconoscere l'esistenza di tutti i popoli ed educarli alla pace e alla fratellanza.